Presidente del Consiglio, al netto della crisi finanziaria mondiale, molta parte dei problemi dell'Italia è nella spesa pubblica e nel debito pubblico. Tutti i Governi sinora hanno tentato di ridurre la spesa con tagli lineari, incidere in modo mirato sulle spese improduttive imporrebbe cambiamenti radicali dell'impianto del bilancio dello Stato, e negli ultimi decenni nessuno finora c'è mai riuscito.

Se le risorse che abbiamo buttato nel debito pubblico le avessimo investite in infrastrutture, innovazione, scuola, università, ricerca scientifica, sicurezza, modernizzazione delle reti, oggi saremmo un Paese più ricco e più forte. forte. Adesso non si può certo abbattere di colpo una così grande montagna di miliardi di debito, ma è doveroso chiedere al Governo quale strategia di medio periodo serva all'Italia, se convengano correzioni virtuose anno dopo anno della spesa pubblica, se convenga puntare sullo sviluppo, se convenga un piano ambizioso di privatizzazioni o un *mix* di tutte queste soluzioni. Vi è una domanda collegata: come possiamo conciliare tutto questo con l'impegno per la riduzione del debito pubblico sino a raggiungere in

due domande su temi strategici della politica economica del nostro Paese. parlando di un tema delicatissimo che sta molto a cuore al mio partito, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ella ha fatto cenno a riforme ed ha innanzitutto confermato il suo impegno e la sua attenzione su questo argomento, e di questo abbiamo preso felicemente atto, ha fatto al contempo cenno a riforme strutturali del nostro sistema di funzionamento dello Stato e delle sue spese, per addivenire positivamente alla soluzione di questo delicatissimo argomento.

andranno ad essere realizzate, fatte salve ovviamente le tematiche sensibili quali la ricerca e i temi che condizionano la sicurezza sociale del nostro Paese e la sua serenità. Nello stesso tempo un altro tema caldo impegna la politica del nostro Paese da tanti anni, forse troppi. Mi riferisco alla dismissione del nostro patrimonio che guardi ad una riduzione sostanziale, direi quasi traumatica, del nostro debito pubblico. Se ne parla da tempo.

di questo progetto - il conferimento di parte del patrimonio disponibile dello Stato ad una società che possa valorizzarlo attraverso cambi di destinazione con conferenze di servizi e quindi in tempi immediati - e la contestuale possibilità di emissione di titoli ed obbligazioni garantiti dal patrimonio immobiliare, che non creino quindi indebitamento pubblico,

per arrivare a questo, vorremmo prima di tutto osservare che, dal terzo trimestre del 2008 fino al primo trimestre di questo anno, in termini percentuali, il debito pubblico italiano è aumentato in realtà in misura minore rispetto a quello di altri Paesi europei come, ad esempio, la Francia, la Germania e l'Austria. c'è da osservare che, in rapporto al PIL, il nostro debito pubblico è tra quelli cresciuti in misura minore dall'inizio della crisi fino al terzo trimestre 2011, momento in cui ci venne imposta la politica di austerità

un pessimo *slogan* mai applicato, abbiamo provveduto a presentare questa mozione, individuando la spesa aggredibile e cercando di impegnare il suo Governo verso un approccio differente da quello attuale. Le chiediamo, quindi, quali sono le misure concrete che il suo Governo vorrà intraprendere, visto che, comunque, si evince dalle sue azioni, fino adesso, che si muoverà comunque nel rispetto del rapporto *deficit*-PIL e, quindi, come vorrà proseguire nella riduzione dell'ammontare del debito pubblico.

di euro, cioè 6 punti di PIL. Questa è l'eredità avvelenata di trent'anni di cattiva politica, che ha scaricato sulle future generazioni un enorme macigno, prosciugandone il futuro. È un macigno che, come lei ben sa, soffoca la nostra economia e impedisce una radicale riduzione della pressione fiscale, condizionando qualsiasi politica pubblica. Ora il *fiscal compact* impone all'Italia di ridurre al 60 per cento il rapporto debito-PIL in vent'anni, ma ma credo che, per rilanciare la nostra economia, abbiamo bisogno di agire molto prima. Allora le chiedo se il suo Governo ha già predisposto un piano straordinario per la riduzione del debito e in che cosa consista questo piano: se comprenda azioni realistiche e credibili di dismissione del patrimonio immobiliare, che, fino ad ora,

comprendere come ella intenda evitare che la privatizzazione di società e aziende venga pagata indebitando le aziende stesse e, quindi, come si possano evitare gli errori compiuti nel passato con tristi casi come Telecom, Alitalia o Aeroporti di Roma, che hanno sostanzialmente impoverito

tocchiamo un tema che sembra laterale rispetto a quello della finanza pubblica, ma che, in effetti, riteniamo sia particolarmente importante. Abbiamo verificato come nel corso degli anni hanno preso sempre più parte, all'interno della finanza pubblica, i proventi derivanti dal gioco d'azzardo (in questo senso, con un crescente che, addirittura, è arrivato al 450 per cento nel corso degli ultimi otto anni). Oggi si parla sostanzialmente, presidente Letta, di un fatturato di ben 76 miliardi di euro, con proventi che derivano allo Stato fino a 14 miliardi di euro. È chiaro che siamo in una situazione di economia in crisi, con famiglie in crisi e, quindi, con finanze familiari in crisi, e ci poniamo una domanda: fino a che punto può essere accettato, anche dal punto di vista proprio morale, che parte dei soldi che servono per dare stabilità alla finanza pubblica derivino da un provento così difficile da giustificare appunto, dal punto di vista morale ed anche economico come il gioco d'azzardo? Noi crediamo che, in questo senso, ci debba essere sicuramente un'attenzione da parte del Governo, e ci interessa anche comprendere quali sono le filosofie che ci saranno nella finanza pubblica nei prossimi anni, tenendo conto, tra l'altro, che si parla anche di proventi che derivano da una situazione tutt'altro che definita. Il gioco d'azzardo, in effetti, ha una parte emersa e una gran parte sommersa, quest'ultima, sommersa come l'evasione fiscale ma in maniera ancora più nefasta, ci preoccupa altrettanto. Sappiamo che il tema è particolarmente avvertito tra tutte le parti politiche. In questo senso, credo ci possano essere anche delle attenzioni che superano gli steccati ideologici. Occorre avere attenzione soprattutto su un aspetto: quello delle *slot machine*, che sono molto diffuse all'interno delle nostre città e nei nostri paesi, ed entrano in maniera subdola anche nelle tasche delle persone. Credo che, in questo senso, sapere dal Governo qual è la sua opinione in merito sarebbe una cosa importante per tutti i cittadini.

venuti agli onori della cronaca, insieme a una pressione fiscale molto forte. Da molte partì si cerca di trovare soluzioni percorrendo strade che sono ormai sperimentate e che in questi ultimi anni non hanno dato un grande frutto, tant'è vero che il PIL scende scende sistematicamente, non recupera, ed è una delle ragioni per le quali il rapporto debito-PIL rimane preoccupante. Noi ci chiediamo, anche in ragione del fatto che sono all'esame del Parlamento provvedimenti come quello in materia di lavoro e come il cosiddetto decreto del fare, se non sia il caso di incominciare a pensare strategie diverse da quelle che invece tradizionalmente sono state perseguite fino ad oggi, coinvolgendo in modo più corale l'intero Paese, grandi parti di questa nostra Italia, a cominciare dalle Regioni. E chiediamo se non si pensa che il patrimonio immobiliare, anziché venderlo, sia molto più utile metterlo a frutto attraverso progetti che rilancino l'economia partendo dalle vocazioni produttive dei luoghi ovvero dalla valorizzazione delle risorse produttive di cui questo Paese è ricco.

Molte aziende, in particolare quelle che operano nel tessile e nella meccanica, a causa dell'eccessivo costo del lavoro nel nostro Paese hanno delocalizzato la produzione in altri Paesi, soprattutto dell'Est europeo. Ciò ha comportato la perdita di moltissimi posti di lavoro, ma ha anche messo in difficoltà molte piccole aziende artigianali collegate a questo tipo di produzione. A ciò si aggiungono altre situazioni, come quelle del settore

viene meno anche la copertura previdenziale ed infortunistica. Anche se mi rendo conto della difficoltà che questo comporta, preso atto dello sforzo che questo Governo sta apprezzabilmente portando avanti a trecentosessanta gradi, le chiedo che cosa intende fare per favorire il rientro delle aziende che hanno portato la loro sede all'estero o vi hanno trasferito rami di attività, non solo per combattere la pesante perdita di posti di lavoro, ma anche la perdita di quel *know how* necessario per lo sviluppo futuro di ambiti economici che erano, e ancora possono essere, strategici per il nostro Paese. Le chiedo inoltre se si intende effettuare un serio censimento

Signor Presidente, presidente Letta, il mio ringraziamento è sentito, anche perché così stempero la mia considerazione nei confronti del Parlamento inglese, e «considerazione» è un termine eufemistico per stemperare quella parola che forse meglio calzerebbe al momento, che è «invidia». E penso di parlare con lei, guardando soltanto lei e non l'intero Governo, così immagino di essere meno in televisione e più in un Parlamento come quello inglese. La considerazione che faccio in proposito, e mi rende facile poterla fare la circostanza che gli altri non l'abbiano fatta, è che sul rapporto *deficit*-PIL come frazione si può lavorare o sul numeratore o sul denominatore. Quanto a lavorare sul numeratore, la richiesta degli altri colleghi mi vede condividere la necessità di chiarimenti in proposito. Mi riferisco al taglio dei rami secchi, delle spese inutili, all'eliminazione della corruzione o a ciò di cui ha parlato nei giorni scorsi, l'emersione del nero favorirebbe non soltanto l'aumento delle entrate, quindi la diminuzione del numeratore, ma anche l'innalzamento del denominatore, dunque con un doppio beneficio rispetto agli altri.

Ma se non si favoriscono le esportazioni italiane, francesi e spagnole, quell'aumento del PIL, che sosterrebbe la possibilità di favorire le esportazioni tedesche, con il tempo verrà a diminuire. L'unica strada è poter intervenire sul cambio dell'euro, e ogni volta che il cambio si è spostato di mezzo punto, le esportazioni italiane sono aumentate del 5

della nostra. Questo dato, che rappresenta un fatto sicuramente positivo per l'Italia, dimostra che il nostro Paese è riuscito a costruire finalmente una situazione strutturale di tenuta dei conti pubblici,

poco, siamo stati in grado di uscire dalla procedura di *deficit* eccessivo aperta dalle autorità europee in modo più semplice di quanto sarebbe accaduto se avessimo avuto invece una crescita del debito maggiore.

Il tema di fondo di questa vicenda è la mancanza di crescita, questione sulla quale il

Quindi, credo che l'elemento essenziale, rispetto anche alle questioni che sono state poste, è dato da una strategia che non può che essere multipla, cioè una strategia giocata innanzitutto sullo spingere sul denominatore. Spingere sul denominatore vuol dire essere in grado di convincere le imprese ad investire e a creare posti di lavoro. Questo sarà uno degli obiettivi principali della legge di stabilità, è stato già uno degli obiettivi del decreto sul lavoro, l'intervento straordinario per la decontribuzione totale e quindi l'incentivo ad assumere giovani, che oggi è operativo. Invito tutti coloro che stanno ascoltando queste mie parole a notare che il nostro Paese oggi ha una condizione di favore fiscale per assumere i giovani che non ha pari

È qui presente il senatore Monti: il Governo del senatore Monti ha introdotto il cosiddetto ACE, cioè uno strumento di incentivazione fiscale che spinge le imprese a capitalizzarsi, ad investire. Credo che questo elemento, legato al fatto che il fisco delle imprese debba essere spinto a guardare lontano e non soltanto e non soltanto al breve, ai vantaggi immediati, sia il secondo grande capitolo. È nostra intenzione caricare su questo tema e cercare di sviluppare fortemente. È ovvio che le politiche per la crescita sono tante e hanno sono tante e hanno a che vedere anche con questioni che devono tenere insieme molti aspetti diversi. Prima veniva citata (e riprendo quello che è stato detto precedentemente dal senatore Ferrara) la questione del contrasto di interessi, perché alla fine questo è il tema, ossia il fatto che il nostro è un Paese nel quale il nero è così alto, il nero è così importante. L'economia nera va combattuta attraverso politiche che devono essere di contrasto, sanzionatorie, ma anche politiche che incentivino, attraverso il contrasto di interessi, all'emersione. Rivendico qui il fatto (ed utilizzo lo spazio che quest'Aula mi consente per parlare ai senatori e ai cittadini italiani) che è in corso un semestre straordinario di incentivazione fiscale come il nostro Paese non ha mai avuto sul tema del cosiddetto ecobonus. È un periodo nel quale il 65 per cento di incentivazione fiscale per ristrutturare casa attraverso tutti gli strumenti di incentivazione e di efficientamento energetico può consentire di far lavorare le imprese, di sistemare per l'appunto le proprie abitazioni in modo tale da avere poi un risparmio energetico, e di fare tutto facendo emergere. Infatti, com'è noto, per avere l'incentivo fiscale bisogna far vedere la ricevuta fiscale, che è l'elemento

di stabilità per il bilancio 2014. Ma è evidente che, accanto alle politiche per far ripartire la crescita del nostro Paese, è necessario continuare sulla linea del rigore, e dico questo sapendo che è una frase che non fa guadagnare molti consensi. Nell'esperienza di ognuno di noi, in famiglia, i propri figli chiedono delle cose per le quali è giusto dire di no, il buon padre di famiglia risponde di no. Penso sia giusto che si sappia che i conti pubblici devono rimanere in ordine, perché il tema del 3 per cento, che è sembrato un tabù, è la condizione che ci consente oggi, per esempio, di avere quelle flessibilità in più che ci permetteranno, nel bilancio del 2014, di inserire investimenti produttivi nuovi che Bruxelles, l'Unione europea ci consentirà proprio perché siamo stati virtuosi. Credo che questo rappresenti un segno importante anche di comprensione, da parte dell'Europa, che non è un rigore, un'austerità cieca: quella sarebbe sbagliata; troppe volte è stata applicata e, giustamente, questo ha portato ad un'immagine pessima dell'Europa. La linea europea sta cambiando, e noi dobbiamo farla cambiare. Il nostro Governo lavora con questo Parlamento e l'Italia è impegnata da tempo per far cambiare la linea Noi dobbiamo dimostrare che la virtù nei conti deve portare dei vantaggi, deve portare cioè la possibilità, come sarà nel bilancio del 2014, di avere una flessibilità e risorse in più sul tema degli investimenti produttivi che saranno infrastrutture, che saranno quindi tagli alle zavorre che il nostro Paese si porta dietro rispetto alla produzione, agli investimenti, al lavoro; tutte questioni che fanno parte di quel pezzo di strategia di medio-lungo termine al quale faceva riferimento il senatore Zanda. Accanto a tutto questo ovviamente la *spending review* è l'elemento essenziale. Noi dobbiamo agire sulle spese improduttive: la tenuta dei conti pubblici sia una tenuta per la quale non si butta via nulla delle risorse pubbliche, per cui ogni risorsa pubblica sappiamo dove va a finire e tutti insieme decidiamo che è giusto che venga spesa. Accanto a questo, però, c'è bisogno poi di operazioni che hanno a che vedere con lo *stock* del debito. Si sono, su questo tema, concentrati molti degli interventi, ad esempio l'intervento della senatrice Lanzillotta e l'intervento del presidente Schifani,

una delle ipotesi a cui ha fatto riferimento il presidente Schifani, che è allo studio: l'ipotesi di una valorizzazione attraverso delle «scatole» che siano in condizione di valorizzare, e poi di allocare, ovviamente nel modo migliore, perché ha ragione la senatrice Lanzillotta - nessuno vuole ripercorrere le strade di privatizzazioni fatte male, che sono state fatte male in altri Paesi e in alcuni casi anche in Italia. La volontà è di valorizzare e di intervenire non soltanto sull'enorme patrimonio pubblico del nostro Paese, ma anche sulle partecipazioni pubbliche nazionali e sulle partecipazioni degli enti locali, sia perché c'è bisogno di efficienza, sia perché c'è bisogno, su questo tema, di allocare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Questa è la somma di tutti gli interventi che faremo. Per quanto riguarda le altre questioni che sono state poste, riprendo quello che ha detto il senatore Candiani: una legge approvata alla fine della scorsa legislatura, la legge n. 189 del 2012 per affrontare il fenomeno della ludopatia, ha

noi in autunno, come ho già detto in quest'Aula l'altro giorno, abbiamo intenzione di approvare, prima, e di applicare, poi (ovviamente sarà questo Parlamento ad approvare, a cambiare e a discutere su questo tema) un grande piano, che si chiamerà «Destinazione Italia», per allargare la possibilità di attrazione degli investimenti in Italia, quindi rendere possibili anche i ritorni cui faceva riferimento il senatore Panizza, si tratta cioè di far sapere che il nostro Paese attrae e vuole attrarre investimenti, perché è attraendo investimenti che poi siamo in grado di dare lavoro. Lo dico molto francamente: se ci sono marchi importanti italiani che trovano investimenti esteri che li rendono più forti sui mercati, io non mi scandalizzo per questo. La parola «italianità» è una parola che oggi va concepita in un'accezione molto più larga. Noi abbiamo bisogno di creare lavoro, di creare occupazione, di creare crescita nel nostro Paese. Se così facciamo, siamo in condizione poi di affrontare anche i temi della finanza pubblica in modo diverso. Infatti - riprendo ancora, in conclusione, quanto detto

Ma la fatica che le nostre famiglie stanno facendo, nonostante il nostro debito sia cresciuto meno degli altri, dimostra che il problema è strutturale: cioè, uno *stock* di debito che ci trasciniamo da tempo e che, come diceva la collega Lanzillotta prima, ci costa ogni anno 90 miliardi di euro soltanto per tenerlo in vita. Una cifra impossibile, che fa sì che ognuno di noi ogni giorno guardi la fatidica e drammatica cifra dei tassi d'interesse, perché se il tasso supera il 5-6 per cento, il

capitoli che già sono legge; una continuità profonda con scelte fatte fino ad oggi; scelte che metteremo nella legge di stabilità; soprattutto, la continuità nella virtù, che è l'unico modo per ottenere risultati di credibilità per i grandi investitori e per creare effettivamente, nel nostro Paese, quella crescita e quella capacità di attrarre investimenti e generare occupazione che rappresentano l'unico modo per uscire dalla crisi.

Il debito pubblico è un problema gravissimo. Le cifre che abbiamo sentito ci dicono quanto pesi anche sullo sviluppo del nostro Paese. La ringrazio in modo particolare per aver sottolineato la necessità che un tema di così grande e consistente dimensione abbia bisogno di una strategia complessiva, nella quale tutti gli elementi abbiano il loro peso: la continuità con la politica virtuosa del rigore;

del Consiglio, mi ritengo soddisfatto, anche se, possibilmente, dell'IMU parleremo in occasione del prossimo *question time*, perché non vi è stato modo di ascoltarla sul tema, ma mi rendo conto che ci sarà tempo, anche perché è un tema delicato, che verosimilmente verrà affrontato in occasione della legge di stabilità.

l'unico gestibile, con intelligenza, con lucidità, ma con determinazione. Credo che occorra mettere a frutto l'esperienza di altre procedure che non hanno dato buoni risultati, mentre cito la norma che ha consentito, in occasione di precedenti finanziarie del precedente Governo, di dismettere parte del patrimonio del demanio militare,

vendita di quei beni. Quindi, il coinvolgimento degli enti locali a che effettivamente questi beni dello Stato possano ottenere una nuova destinazione, e quindi una valorizzazione, con un interesse dell'ente locale, che naturalmente non può non tenere a mente l'interesse pubblico, e pertanto l'interesse della pianificazione urbanistica. Quindi, cambi sì, ma in sintonia con la gestione del patrimonio e l'indirizzo urbanistico, lo sviluppo delle città.

che la riduzione del debito dovrà essere uno dei temi su cui il suo Governo e la sua maggioranza dovranno più impegnarsi. credo che il tema che abbiamo toccato necessiti assolutamente di approfondimento e certamente di ulteriori provvedimenti di legge. Come spesso accade, il il male si presenta sempre con una veste banale, come un seme molto piccolo, che poi cresce e penetra con radici profonde. È il caso del gioco d'azzardo, che nelle nostre comunità è entrato in maniera molto profonda. Chi, come me, è stato sindaco sa quanto le comunità siano in difficoltà per queste realtà. Presidente, abbiamo presentato un disegno di legge e ve ne sono già altri depositati agli atti del Senato: portiamo in discussione una moratoria e diamo un esempio, a partire dalla riduzione delle aspettative di gettito dal gioco d'azzardo.

troviamo sempre ragioni d'intesa sull'analisi dei problemi che abbiamo di fronte. Del resto, SEL non sta facendo un'opposizione

ad una discussione e produrre un piano pluriennale straordinario, organicamente gestito per lo sviluppo e l'occupazione, senza tagliare fuori nessuno, senza produrre in modo sistematico decreti-legge che poi subisce questo Parlamento, ma soprattutto subiscono gli enti locali, le Regioni e i cittadini. Faccia partecipare meglio tutti alla costruzione del futuro. che questa pratica sia quella che il Governo si vuole dare. Signor Presidente, apprezzo la grande concretezza, ma anche il senso del rigore del presidente Letta, peraltro caratteristiche che lo contraddistinguono sempre quando interviene in quest'Aula. Se le ho rivolto oggi questa domanda è perché la situazione purtroppo sta peggiorando e le politiche promozionali portate avanti da Paesi noi confinanti (forse noi viviamo peggio di altri questa situazione) stanno purtroppo producendo degli effetti, perché evidentemente la differenza

lunga tradizione di lavoro che contraddistingue il nostro Paese, ha sempre caratterizzato l'Italia. Mi auguro che oggi l'eccessivo carico fiscale e l'eccessivo costo del lavoro non vanifichino una tradizione lavorativa e un prestigio internazionale conquistato in tanti anni di lavoro duro e, quindi, non vanifichino i risultati che le nostre aziende hanno ottenuto sui mercati mondiali.

ed esporta il 50 per cento di quanto esporta l'Europa all'estero, ma se l'Europa non cresce, il rimanente 50 per cento che la Germania esporta in Europa, non avrà più a chi esportarlo.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, non sfugge a nessuno che la preoccupazione più grande delle famiglie italiane oggi è il lavoro dei propri figli. È la prima volta, nella storia delle generazioni, che le ragazze e i ragazzi rischiano di avere un futuro più incerto delle madri e dei padri. La vita lavorativa stessa è diventata un rischio: con le numerose crisi aziendali ci sono tante lavoratrici e lavoratori cinquantenni che vedono in pericolo il loro futuro. Ma noi del futuro abbiamo tanto bisogno, e di fiducia. Lei, signor Presidente, ieri ha dichiarato che non possiamo fermarci a queste difficoltà, ma dobbiamo avere obiettivi di risorse e obiettivi di visione. Nella raccomandazione del Consiglio europeo sull'istituzione di un garanzia per i giovani, si ricorda che spesso i giovani non dispongono di esperienza professionale, hanno un grado di istruzione o una formazione non sufficiente e non adeguata al mercato del lavoro, hanno un accesso ridotto a risorse finanziarie e condizioni di lavoro precario. Nel decreto che lei ha ricordato prima, signor Presidente, e che è in discussione in quest'Aula, ci sono misure che si propongono di rafforzare la rete dei servizi

Nello stesso tempo è necessario trovare risorse sufficienti per coprire le esigenze della cassa integrazione in deroga. Le chiedo, allora, signor Presidente, come il Governo intenda affrontare il tema dell'integrazione vera e solida tra politiche attive e passive del lavoro, per consentire alle nostre cittadine e cittadini di essere accompagnati in tutto l'arco della vita: dalle aule scolastiche, all'accesso al lavoro, alla formazione permanente, al sostegno al reddito nei momenti di difficoltà. chiedo se non sia giunto il momento di attuare politiche per la crescita - da lei giustamente ricordata prima - accanto a politiche di cura dell'occupabilità della forza lavoro

*(PdL)*. Presidente Letta, alcune proposte utili per rilanciare l'occupazione, soprattutto tra i giovani, sono contenute nel cosiddetto decreto lavoro all'esame del Senato. Confido nella buona volontà di tutti noi per produrre un testo di qualità. Mi preme però chiederle qualcosa di più complessivamente strategico, perché il lavoro - lo ricordava lei stesso nella sua prima risposta - non è una variabile indipendente, non è un comparto a sé stante, ma è un tassello fondamentale della politica economica di un Paese. Gli studi OCSE e INPS, resi recentemente pubblici, hanno riclassificato il lavoro come emergenza nazionale, specie nel confronto con l'Europa. Nell'ultimo anno il mercato del lavoro, in entrata come in uscita, continua ad essere troppo rigido, ulteriormente appesantito da alcuni cascami della cosiddetta legge Fornero. Il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il 12,2 per cento e le stime per il 2014 indicano purtroppo un ulteriore incremento. Le maggiori fragilità sono tra i giovani, i lavoratori di mezza età e i lavoratori scarsamente qualificati. Il Popolo della Libertà è convinto che la ripresa dell'occupazione possa essere supportata dal decreto lavoro, ma è convinto altresì che il Governo debba impegnarsi strategicamente verso l'obiettivo della riduzione complessiva della pressione fiscale - abolizione dell'IMU sulla prima casa, non aumento dell'IVA, taglio del cuneo fiscale - e verso misure specifiche di incentivazione, semplificazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro. Plaudiamo anche noi agli accordi in sede europea per lo *Youth Guarantee*, come alle opportunità del progetto «*New deal for Europe*»; tuttavia ci preoccupa, ad esempio, la scarsa pervasività percentuale dei nostri centri per l'impiego rispetto alle analoghe strutture europee. Tutto ciò premesso, presidente Letta, pongo la seguente domanda: quali forme di semplificazione, flessibilizzazione e riduzione della pressione fiscale il Governo intende mettere in campo per incrementare l'occupazione e la ricerca di lavoro, soprattutto dei giovani e di quanti siano già entrati o stiano entrando nel tunnel tunnel della disoccupazione? Magari si pensa ad una formula sul modello dell'EXPO 2015? Come intende il Governo potenziare e rendere più efficienti i centri per l'impiego, anche per incidere sul numero montante dei nuovi disoccupati e dei giovani NEET, che né studiano né si formano né cercano lavoro?

BENCINI *(M5S)*. Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi, le imprese italiane si trovano in una grave crisi dovuta alla globalizzazione che ha colpito quasi tutti i settori produttivi e in uno svantaggio competitivo nel quale vertono rispetto alla concorrenza di aziende straniere, con conseguente impoverimento dell'occupazione nel nostro Paese.

su una platea potenziale di circa 3 milioni di persone. I vincoli di finanziamento consentono di incentivare l'assunzione al massimo di 50.000 giovani lavoratori all'anno, per un totale di circa 100.000 lavoratori. Nel nostro Paese ci sono ben 160 aziende in grave crisi industriale, come Ilva, Lucchini, Berco e molte altre; vi sono poi altre aziende che la crisi la creano scegliendo di delocalizzarsi. La delocalizzazione delle imprese italiane è stata prevalentemente del tipo *low cost seeking* ovvero fondata sulla ricerca della riduzione del costo della manodopera e concentrata in settori produttivi ad alto valore aggiunto. Oltre alla grande industria, quasi trent'anni fa è iniziata la delocalizzazione della piccola e media industria della Toscana (ad esempio, pellami, calzature, stoffe di medio livello). anni dopo, ma più massicciamente, ha iniziato l'industria del Veneto, che aveva già esperienza *in loco* di internazionalizzazione della produzione, con il ricorso all'abbondante manodopera frontaliera dell'attuale Slovenia con esso confinante. La ricerca del minor costo del lavoro *tout court* è invece spinta non dagli alti livelli salariali dei lavoratori italiani, ma dal costo complessivo del lavoro gravato a carico dell'impresa quasi di un altro 50 per cento per i contributi parafiscali, il cui importo dovrebbe garantire l'alto livello di *welfare* in Italia: assistenza medico-ospedaliera gratuita per tutti, assicurazione pubblica per gli infortuni sul lavoro, pensioni, indennità di fine rapporto e 30 giorni di ferie l'anno. Alla luce di tutto ciò, il Movimento 5 Stelle domanda in che modo il Governo può arginare questa migrazione produttiva, evitare la svendita del nostro *know-how* al fine di preservare la nostra capacità imprenditoriale e quindi garantire posti di lavoro, oltre che riuscire a crearne di nuovi.

siamo consapevoli di quanto sia importante per il Governo il tema della disoccupazione, soprattutto giovanile. Vogliamo però attirare la sua attenzione anche sulle raccomandazioni dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di mercato del lavoro, che sono costanti e sono già state oggetto di precedenti interventi legislativi. In questo contesto le chiediamo se non ritenga opportuno che vengano messe in cantiere, per cogliere le opportunità di ripresa che seppur timidamente si affacciano, a cominciare dall'Expo 2015, misure ulteriori volte a compensare la straordinaria incertezza che caratterizza il quadro in cui le imprese sono costrette ad operare, riducendo il disincentivo normativo all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Pensiamo, in particolare, alla possibilità di consentire, almeno fino alla fine del 2015, l'assunzione a tempo indeterminato con minori costi e minori vincoli e l'eventuale scioglimento del rapporto, almeno nel triennio iniziale, e nel periodo successivo con una protezione della stabilità del rapporto crescente al crescere dell'anzianità di servizio del lavoratore.

Dobbiamo renderci conto che, cittadini italiani e immigrati regolari, siamo tutti sulla stessa barca: siamo in recessione, non c'è lavoro per nessuno.

e onestamente avere una valutazione d'impatto dal punto di vista lavorativo per i giovani è molto arduo, perché ho l'impressione che ne avrà veramente molto poco.

anche a lei: è la questione su cui tutti i cittadini, dovunque andiamo, ci chiedono notizie, informazioni; vogliono sapere cosa ne sarà di loro se perdono il posto di lavoro magari tra uno o due anni. Non riguarda soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche piccoli imprenditori

di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parti di essi, il trattamento straordinario d'integrazione salariale per crisi aziendale

In particolare, nel caso di Whirlpool (che lei conosce benissimo perché gliene hanno parlato anche al Festival dell'economia), tutte le istituzioni locali e anche la nostra comunità sono particolarmente preoccupate per le conseguenze negative che ha sull'indotto di tutte le aziende artigianali che con la Whirlpool lavoravano. locali si stanno muovendo bene di concerto con le parti sociali per fare in modo che lo stabilimento non chiuda, ma trovi una nuova proprietà; questa soluzione, però, ha bisogno dei suoi tempi, nei quali è importante tutelare la comunità dei lavoratori che oggi è fortemente preoccupata. Le chiedo pertanto se il Fondo per l'occupazione dispone di risorse sufficienti a finanziare le proroghe dei programmi di cassa integrazione previsti dalla norma che ho richiamato o se, in una logica di aiuto in una fase così difficile per la tenuta economica e sociale del Paese, non si intenda rifinanziarlo per la gestione dei recenti gravi casi di chiusura di stabilimenti come quelli che ho appena citato e fra i quali le ricordo, in particolare, la Whirlpool di Trento. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, l'attuale fase di grave crisi occupazionale, specialmente giovanile (come hanno detto molti miei colleghi), che attraversa il Paese, è conseguenza della più ampia sfavorevole congiuntura economica e non trova certamente giovamento dalla riforma del sistema pensionistico realizzato con la legge Fornero. rilevata l'indubbia importanza che rivestono sul fronte occupazionale determinati settori, sia pubblici che privati, come quello rappresentato dalle piccole e medie imprese, che sono il vero motore dell'Italia, ma anche quello sanitario, in cui l'accesso alla professione per i giovani medici,

Si chiede al Presidente del Consiglio se il Governo non ritenga opportuno intavolare una riflessione sull'opportunità di prevedere una sorta di scivolo per gli addetti in sovrannumero a quei servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale ormai esternalizzati e per i professionisti del settore che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi pre-riforma Fornero e facciano facciano richiesta di pensionamento, immaginando di procedere ad una assunzione di personale medico, sanitario, paramedico per ogni quattro collocamenti a riposo del personale di cui sopra. Si chiede altresì se l'Esecutivo non ritenga di procedere con lo sblocco del Patto di stabilità in quelle Regioni colpite negli ultimi due anni da fenomeni sismici significativi, così che le relative amministrazioni possano provvedere con maggiore velocità e capacità di spesa alla ricostruzione, agevolando anche la ripresa dell'attività in quelle aziende la cui importanza è vitale per i rispettivi per i rispettivi territori, specialmente sotto il profilo occupazionale. Ricostruzione e risposta occupazionale, ad esempio, nella mia Lunigiana e nella vicina Garfagnana - che lei, perfettamente - sarebbero attuabili sottraendo ai vincoli del Patto di stabilità esclusivamente le risorse che la Regione Toscana si è già impegnata a destinare per far fronte all'emergenza postsismica. quindi un emendamento da inserire in un decreto e il problema sarebbe risolto per tutte le zone che sono state colpite da fenomeni sismici rilevanti.

fa parte sicuramente del cuore della nostra missione, sicuramente comune dalle parole che ho ascoltato fino adesso. È un tema particolarmente caldo, perché mai come negli ultimi anni la crescita della disoccupazione, e della disoccupazione giovanile ancora di più, ha colpito il nostro Paese. tutti sappiamo che abbiamo una missione: questa missione è lavorare perché l'Italia riprenda il cammino dell'occupazione e della creazione di lavoro. Quale lavoro? Molti interventi hanno toccato proprio il tema dell'attualità del lavoro, e su questo voglio insistere, su un punto che ritengo essenziale. Tutto ciò che abbiamo svolto fino adesso, nei novanta giorni

Lo voglio dire con forza perché non contano solo le parole, anche se pronunciate in quest'Aula, dove le parole pesano e contano di più: contano i fatti. Questo Governo ha fatto una scelta. Questo Governo ha scelto di incentivare il lavoro a tempo indeterminato, perché riteniamo che sia fondamentale nel nostro Paese dare alle imprese e ai lavoratori la possibilità di stabilizzare rapporti di lavoro il più lungo possibili, serve alle imprese e serve al lavoratore: serve alle imprese, che investono sulla professionalità del lavoratore, e serve naturalmente al lavoratore, che si crea una prospettiva di vita, un progetto di vita molto particolare e di lungo periodo.

hanno fatto due giorni fa. È una scelta molto importante innanzitutto perché l'hanno fatta insieme e io ho intenzione di lavorare insieme alle parti sociali, lo ritengo fondamentale. Ho incontrato ieri i sindacati e incontrerò nei prossimi giorni i rappresentanti del mondo delle imprese. Ho intenzione di lavorare con tutte le mie forze perché ci sia la corresponsabilità e la capacità di scegliere insieme, fermo restando che poi sarà quest'Aula, a cui il Governo proporrà le scelte che ritiene più importanti e migliori da fare,

(su cui, con i sindacati nazionali, cercheremo di lavorare, perché quell'esperienza positiva possa essere un'esperienza positiva che si allarga), ma anche su altri temi. L'Expo sarà una grandissima opportunità per l'Italia: sarà un'opportunità per creare lavoro e investimenti positivi e per dotare di infrastrutture un'area del nostro Paese che ne ha terribilmente bisogno. Il tema essenziale dell'Expo è un tema rispetto al quale la possibilità di agganciare la crescita lì è legata a cosa facciamo adesso. E cosa facciamo adesso vuol dire tante cose: vuol dire - ovviamente - fare scelte che diano investimenti, che diano lavoro e - naturalmente - che diano legalità. All'Expo ho intenzione di legare normative nazionali che rafforzino quegli elementi di tutela e di legalità che sono essenziali perché questo carico

disillusione, di delusione o di critica perché una parte significativa delle risorse è stata caricata sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile. Lo so: so che i disoccupati sono di tutte le età,

cioè che hanno perso il lavoro e hanno l'ultima parte di protezione sociale. Abbiamo inserito un provvedimento che incentiva le imprese ad assumere quei lavoratori, che evidentemente non sono lavoratori giovani perché si tratta di persone che già lavoravano e che hanno perso il loro lavoro. L'impresa che li assume avrà i vantaggi dell'ASpI per tutto il periodo che rimane. Credo che questo sia un segnale molto forte. Lo dico perché prima la senatrice Bencini ha giustamente citato la difficoltà dei lavoratori di tutte le età e anche il fatto che i lavoratori che hanno una certa età fanno poi più fatica a ricollocarsi. c'è uno strumento, ed è uno strumento che io voglio esaltare perché dimostra che l'attenzione a non lasciare nessuno indietro è un atteggiamento di cui noi siamo assolutamente convinti.

Il rappresentante della Lega Nord ha citato la questione dei flussi e quella dei lavoratori extracomunitari. Noi abbiamo un sistema normativo fatto a fisarmonica: voglio dirlo, perché credo sia importante che si sappia. È un sistema per il quale, nel momento in cui cresce la disoccupazione dei lavoratori stranieri più di quella dei lavoratori italiani, si interrompono i decreti flussi.

stata applicata anche in questa situazione. Ovviamente spero e mi auguro ardentemente che cali la disoccupazione sia per i lavoratori italiani sia per quelli stranieri, perché abbiamo fortemente bisogno che su molti lavori ci sia un rilancio e una possibilità.

che è stata ovviamente al centro dell'ultimo Consiglio europeo. Come sappiamo, l'ultimo Consiglio europeo ha affrontato questo tema: nella riunione che abbiamo svolto a Berlino, alla quale ho partecipato insieme al ministro Giovannini, insieme ai rappresentanti di tutti gli altri Paesi europei, la questione dei servizi per per l'impiego è stata centrale. Il nostro Paese ha una carenza sul tema dei servizi per l'impiego; è una carenza assolutamente evidente, della quale bisogna prendere atto. Non abbiamo un servizio per l'impiego all'altezza della sfida della disoccupazione attuale; non abbiamo un investimento pubblico sufficiente; facciamo fatica su questo tema. È una fatica della quale credo

uno degli elementi essenziali è l'Unità di missione, a partire dalla quale si comincerà a lavorare. L'Unità di missione si insedierà martedì

alle esperienze di successo che ci sono negli altri Paesi europei. La riforma strutturale del servizio per l'impiego è una delle principali riforme strutturali che abbiamo davanti. Saremo obbligati anche dal tema della «Garanzia per i giovani», perché la *Youth Guarantee* è un elemento che obbligherà il nostro Paese a dare risposte e a legare la domanda all'offerta, in particolare dopo il percorso formativo, con modalità che fino ad oggi non si sono mai applicate. lo stesso decreto, come sapete, dà il via finalmente alla costituzione di una grande banca dati, che sarà essenziale per legare insieme domanda e offerta. Credo che questo sia il tema sul quale l'impegno dei prossimi giorni sarà rivolto a cercare cercare di riprendere il tempo perduto di far sì che domanda e offerta si incontrino. Siamo ovviamente prontissimi e attentissimi - lo dico rispetto agli argomenti che il senatore Susta poneva prima

assente. Voglio citare la carta per l'inclusione sociale: è una novità importante che dimostra la volontà di questo Governo di affrontare il tema della povertà estrema, povertà estrema, una delle grandi sfide della democrazia, perché essa non ha normalmente rappresentanza: la povertà estrema, nella gran parte dei casi, non vota. La povertà estrema è diffusa nel nostro Paese, c'è, ed è necessario dare risposte. La carta per l'inclusione sociale è una prima risposta: dico prima risposta perché interviene per il Mezzogiorno e per le grandi città metropolitane. La carta per l'inclusione sociale dà una prima risposta sulla cui falsariga dovremo lavorare, ma la voglio citare in questa sede perché attorno al tema della disoccupazione sappiamo tutti che, molto spesso, il passo tra la disoccupazione e i limiti di povertà è uno di quelli che deve angosciare coloro che siedono in questi e negli altri banchi di quest'Aula, perché il nostro Paese, a seguito di questa crisi, sta vivendo un'estensione di difficoltà familiari e territoriali che, in particolare in alcune aree del nostro Paese, stanno diventando insostenibili. Questo è il motivo per il quale affrontare questi temi con la determinazione e soprattutto soprattutto passo passo, come dicevo prima, è una grandissima priorità; è ciò che stiamo facendo, è soprattutto ciò che insieme a voi vogliamo fare ancora di più.

noi stiamo convertendo in legge il decreto-legge n. 76 del Governo e non c'è da interpretare: ci sono gli incentivi per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato; quindi questo è un fatto. In secondo luogo, non possiamo affrontare le politiche del lavoro senza appunto una prospettiva di visione futura e il tema della domanda-offerta domanda-offerta di lavoro è cruciale perché dobbiamo rafforzare la forza lavoro che abbiamo e quella che avremo. Anche in questo caso è un tema di grande democrazia perché attiene alle pari opportunità di accesso per tutti, chi può e chi non può, al lavoro e risponde alla domanda:

edificante, in una fase in cui non è facile essere costruttivi, e questo lo apprezziamo molto. Pertanto anch'io mi ritengo soddisfatta. Certamente dovremo lavorare ancora molto, dovremo lavorare insieme; questo è il senso della nostra continua presenza e del nostro continuo apporto sui provvedimenti. In particolare mi fa piacere che ella abbia voluto stigmatizzare e segnalare con particolare attenzione il tema del felice e fortunato negoziato Expo 2015. È vero che proprio su quei presupposti possiamo raggiungere ed acquisire quell'esigenza di semplificazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro senza la quale, ahimè, l'unità di misura della ricchezza nel nostro Paese, cioè l'impresa... *(Il microfono senatrice Bernini. BERNINI *(PdL)*. Sappiamo che il lavoro non si crea per decreto, anche il lavoro a tempo indeterminato, e che da sempre le catene dell'impresa stanno nelle carte dei regolamenti inutili.

sgravare dei costi del lavoratore. e poi ovviamente hanno fatto il salto ma non ce l'hanno fatta a saltare e sono rimasti completamente nel vuoto: questi sono proprio fuori dal circuito in questo momento. Ancora, vorrei dire che per creare lavoro è

il costo d'impresa sia sicuramente minore. Ancora, lei ha detto che nessuno deve rimanere indietro: in questo momento in Italia sono circa sei milioni le persone che sono rimaste indietro e che hanno un *gap* abbastanza importante rispetto a quelli che sono avanti.

quello che lei ha voluto dire, cioè che il Governo è fortemente impegnato in riforme strutturali, vorremmo sottolineare tre aspetti. Il primo è quello della formazione professionale, che va comunque rivista di concerto con le Regioni e con gli enti locali. revisione degli ammortizzatori sociali: non possiamo pensare che sia solo la cassa integrazione risolutiva dei bisogni che ci troviamo di fronte. Il terzo è che comunque la questione del mercato lavoro deve essere vista da parte di chi è il vero datore di lavoro: la politica può aiutare a rimuovere gli ostacoli che ci sono alle assunzioni, ma oggi bisogna mettere in condizione soprattutto le imprese di affrontare le emergenze che ci sono, anche per poter reggere la concorrenza sui mercati mondiali. Da questo punto di vista, assolutamente necessario che ci poniamo il problema della centralità di chi davvero deve dare il lavoro oggi, che è il sistema delle imprese: ma le sue parole sono

quartieri-ghetto, dove ci sono campi rom, con situazioni al limite del degrado sociale. Si è parlato di Expo. Ebbene dobbiamo evitare che accada quello che è successo a Shangai qualche anno fa (chi è stato a Shangai lo può dire tranquillamente):

Sul discorso della carta per l'inclusione sociale, anche se non era una mia domanda, le chiedo, Presidente, prima di iniziare questo tipo di operazione, magari di

tolto il campo rom per far vedere che andava tutto bene. Questa è l'Italietta. Spero che lei non sia a favore dell'Italietta! [DE Presidente Letta, devo registrare che sulla questione degli esodati e sulle idee del Governo su come intervenire in modo strutturale per rivedere i meccanismi che producono ogni giorno lo stesso fenomeno della riforma Fornero lei è stato abbastanza evasivo, e me ne dispiaccio.

facendo in alcune forme, ma anche a dare un profondo impulso sulle questioni dell'innovazione (che in parte sono toccate con le *start up*):

Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per la sua risposta, che naturalmente ho apprezzato e della quale mi ritengo soddisfatto; la ringrazio soprattutto perché conferma la volontà di trovare sempre, non solo la collaborazione, ma anche l'intesa con le istituzioni locali, e credo che questo sia il modo migliore per operare. Le confermo che, nella nostra autonomia responsabile, si sta facendo tutto il possibile per mettere in campo ogni strumento che possa risolvere questa situazione difficile. Sono molto soddisfatto che in questi giorni siano stati raggiunti importanti accordi con le aziende e le forze sociali, che credo

si sarebbe fatto un semplice bagno. La legge Fornero ha portato disoccupazione perché è stata varata bruscamente; si è infatti passati da una quota 96-97 a una quota 109-112,

un neurochirurgo non si può sostituire con un cuoco. Abbiamo bisogno di aumentare quel *turnover* di alta specializzazione, nell'interesse del Servizio sanitario nazionale e della salute pubblica. Credo che la rivisitazione in questo senso della legge Fornero riporterà

La seduta è tolta